Comunico che, in data 26 maggio 2008, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» Onorevoli colleghi, è stata presentata dal prescritto numero di senatori una mozione con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sulla messa al bando delle bombe a grappolo. In vista dell'imminente conclusione della Conferenza internazionale di Dublino per la messa al bando delle bombe a grappolo, la mozione, insieme ad altre eventualmente presentate sullo stesso tema, sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea nel corso di questa settimana, a partire da domani, a conclusione della discussione dei decreti-legge calendarizzati. Dopo l'illustrazione, i Gruppi potranno intervenire nel dibattito per venti minuti ciascuno, comprensivi dei tempi della discussione generale e delle dichiarazioni di voto. Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in Libano». Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione 10 minuti.

onorevoli senatori, come voi sapete, l'accordo che è stato raggiunto a Doha la settimana scorsa pone fine ad una crisi molto complessa che era iniziata nel novembre del 2006 con le dimissioni dell'Esecutivo del primo ministro Siniora, dei cinque Ministri di confessione sciita e del titolare dell'ambiente cristiano vicino all'allora presidente filo-siriano Lahoud. Ciò ha aperto un'evidente crisi politica che ha paralizzato per 18 mesi il Libano, spaccando il Paese in due campi fortemente contrapposti.

ritenendo che fosse venuta meno la presenza proporzionale nel Consiglio dei ministri delle principali confessioni religiose presenti nel Paese e, dall'altro, invece, le forze della maggioranza che hanno considerato sempre l'Esecutivo Siniora legittimo, come d'altronde hanno fatto i principali partner internazionali che hanno avuto relazioni formali, diplomatiche e di cooperazione in questo periodo con il Governo Siniora, Siniora, non ritenendo - questa era l'opinione del primo ministro uscente Siniora - che fosse a loro imputabile istituzionalmente la fuoriuscita dei Ministri sciiti. sciiti. Tra l'altro, il premier Siniora non aveva accettato formalmente le dimissioni di quei sei Ministri, che si trovavano quindi nella posizione di essere dimissionari, ma ancora formalmente in carica, cioè di svolgere sia pure indirettamente alcune delle loro funzioni. Il problema principale era l'assoluta sfiducia tra le varie componenti, aggravata da uno stillicidio davvero orribile di attentati che hanno colpito, tra l'altro, esponenti del Parlamento. Ciò non ha consentito per un lungo periodo un accordo sui tre punti principali: l'elezione di un Presidente della Repubblica (carica vacante dallo scorso 24 novembre); la formazione di un Governo di unità nazionale e l'adozione di una nuova e condivisa legge elettorale.

Siniora. All'inizio del mese di maggio, la decisione che ha in qualche modo smosso questa situazione apparentemente di equilibrio (ma di equilibrio negativo, ovviamente) è stata la decisione di rimozione del generale Shukair, capo dei Servizi di sicurezza dell'aeroporto di Beirut, persona vicina ad Hezbollah, di confessione sciita, che è stato rimosso con l'accusa di avere compiuto attività non consentite di monitoraggio dello scalo aeroportuale di Beirut.

sette giorni di scontri, 72 morti, 242 feriti. In questa situazione la Lega araba (e in particolare un autorevole membro della Lega stessa, cioè l'Egitto) ha promosso una riunione straordinaria che ha condotto ad una missione a Beirut di un comitato della Lega araba guidato suo segretario generale Amr Moussa, dal Primo ministro del Qatar e composto da otto Ministri degli esteri di Paesi arabi. In tale ambito ha inizio la recente azione

mi sono trovato nella situazione, ovviamente consapevole e voluta, di avviare una serie di contatti un contributo del Governo italiano ad un'azione di raccordo e di forte sostegno all'iniziativa diplomatica della Lega araba, che mi è sembrata dal primo minuto iniziativa ragionevole e positiva. Tale azione di raccordo è stata condotta insieme dal Governo italiano, dagli Stati Uniti d'America, dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito - quindi, da quattro partner europei - e dagli Stati uniti d'America. Ovviamente, ho sentito il bisogno di un contatto immediato con il primo ministro Siniora e con il presidente del Parlamento Berri, leader di Amal. Ad entrambi ho in primo luogo ribadito, già il nove maggio, la vicinanza del Governo italiano in quel momento molto critico, vicinanza evidentemente unita alla condanna, altrettanto chiara, per l'inaccettabile ondata di violenza in corso che si manifestava con le strade bloccate, i blocchi stradali e le milizie di Hezbollah che avevano preso possesso di alcuni quartieri di Beirut. Abbiamo concordato in quelle ore un ulteriore incontro, una conferenza telefonica allargata del gruppo da noi definito di «Amici del Libano», un gruppo di Ministri degli esteri di circa 15 Paesi. hanno ovviamente partecipato i Ministri europei dei Paesi citati in precedenza, molti Ministri degli esteri di Paesi della Lega araba, gli Stati Uniti e - in collegamento - anche il segretario generale dell'ONU Ban Ki-Moon. conferenza telefonica il 10 maggio abbiamo concordato che, sostanzialmente, una missione come quella della Lega araba meritava il sostegno assoluto e incondizionato perché fondata sull'obiettivo dichiarato di far raggiungere un accordo alle forze politiche libanesi. Tale accordo vi è stato, dopo un invito concorde dei partiti politici a Beirut alla delegazione della Lega araba, che aveva il suggello dei 15 Paesi che formano il gruppo degli «Amici del Libano» e che ha posto le basi per i negoziati di Doha. L'impegno, anche personale, dell'Emiro del Qatar è stato determinante: determinante: egli ha condotto un'azione di persuasione per condurre a Doha la missione e tutte le delegazioni interessate che, nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso, hanno raggiunto un accordo. un accordo. Si tratta di un accordo basato su alcuni punti: l'elezione alla Presidenza della Repubblica, avvenuta domenica scorsa - ed io sono stato presente

da 30 Ministri, di cui 16 per la maggioranza, 11 per l'opposizione e 3 che saranno designati dal presidente Suleiman; infine, terzo punto, il ritornodella legge elettorale

a non ricorrere all'uso della forza e a non usare le armi all'interno del territorio libanese, con ovvia eccezione della sola autorità legittimata, cioè l'esercito libanese e le relative forze di polizia, nonché l'impegno politico ad avviare subito, in parallelo, un dialogo per rafforzare quella che è stata definita nell'accordo autorità dello Stato libanese. Chi ha ottenuto cosa? L'opposizione

mezz'ora dopo la sua elezione - debbo dire che l'Italia è stato il primo Paese con cui il presidente Sleiman ha accettato un incontro bilaterale - ha detto sarà formato nelle prossime settimane e quindi in tempi molto rapidi.

La richiesta dell'opposizione era anche quella di avere un sostanziale potere di veto sui provvedimenti di riforma costituzionale ed é stato innalzato il *quorum*, in modo da consentire che le riforme costituzionali vengano adottate - il che mi sembra logico - anche con il contributo necessario dell'opposizione. La comunità cristiana, quindi l'altra parte, ha ottenuto un successo altrettanto importante perché, se analizziamo la legge elettorale del 1960 che è quella secondo la quale si voterà nella primavera del 2009 per le elezioni politiche, il Partito cristiano potrebbe recuperare in modo significativo la sua influenza dato che la distribuzione dei collegi sulla base delle piccole circoscrizioni - il nuovo sistema elettorale crea più circoscrizioni, ma con territorio più limitato permetterà presumibilmente all'elettorato cristiano di eleggere i propri parlamentari con una maggiore autonomia rispetto al condizionamento forte sul terreno che la legge del 2000 conferisce alle altre due comunità, quella sciita e quella sunnita. È chiaro che le forze della maggioranza sunnita hanno espresso soddisfazione perché

molti di voi lo sapranno, ma domenica sera il Ministro degli esteri di Damasco era presente ufficialmente, come capo della delegazione siriana, ad assistere all'elezione del

che considero una *condicio* *sine qua non* per la stabilizzazione istituzionale del Libano e per il suo consolidamento, cioè la necessità di attuare pienamente la risoluzione n. del Consiglio di sicurezza che prevede il disarmo di tutte le milizie, innanzitutto della milizia di Hezbollah. Questo è un punto esplicitamente richiamato nell'accordo di Doha, che definisco una *condicio* *sine qua non* perché, come ha detto il presidente Sleiman nel suo intervento, se non ci sarà un parallelo smantellamento delle milizie e un consolidamento di un nuovo esercito libanese con mezzi, strutture e professionalità il consolidamento istituzionale del Libano non ci sarà.

Il partito di Hezbollah, che probabilmente avrà ministri nel prossimo Governo, evidentemente è di fronte ad una sfida: o assumere una corresponsabilità per attuare in pieno l'accordo di Doha, non soltanto le parti preferite, quindi quindi partecipare al consolidamento del Libano, oppure mantenere un atteggiamento di distinzione tra parti dell'accordo che si preferiscono e parti che si vogliono nascondere. Spero che ciò non accada, anche se la percezione che ho avuto, per quanto mi hanno detto gli interlocutori libanesi, è che dopo il conflitto del 2006 Hezbollah ha perso le simpatie di una larga parte

è stato visto attaccare con le armi altri libanesi determinando un impatto molto forte nella percezione della popolazione civile libanese a scapito dell'immagine delle milizie. La seconda incognita è il contesto regionale, particolare l'evoluzione dei contatti tra Libano, Siria ed Israele. In prospettiva vedo una possibilità di normalizzazione tra Libano e Siria. Il regime di Damasco ha apprezzato, come vi ho detto, partecipando con la presenza del Ministro degli esteri - dunque, una presenza di alto livello che non si era mai vista in una cerimonia così formale - all'elezione del presidente Sleiman e ha ribadito di attribuire la più grande importanza al rispetto della sovranità libanese. Si tratta di un punto chiave: come ha detto il presidente Sleiman - e io lo sottoscrivo non vi potrà essere normalizzazione se non basata su due punti chiave, l'autonomia e l'indipendenza della nazione libanese rispetto ad ogni altra nazione vicina. quindi che il principio dell'autonomia e dell'indipendenza sarà la chiave per avviare un negoziato sulla normalizzazione, ivi compresa la demarcazione delle frontiere, che, come sapete, è un tema ancora aperto.

e in cui evidentemente l'attività delle milizie sul territorio continua. Sapete perfettamente che le milizie di Hezbollah hanno preso della loro autodefinita resistenza anti-israeliana la questione mai risolta di un territorio piccolo, ma simbolicamente importante, quello delle fattorie di Shebaa, controllato dall'esercito israeliano e conteso, come sapete, tra Libano, Siria e lo stesso Israele. C'è però un aspetto

per la restituzione ad Israele di due soldati israeliani presi prigionieri durante il conflitto del 2006. Auspico naturalmente con tutto il cuore che tali contatti portino davvero alla liberazione dei soldati israeliani

caselle, questi tasselli, procederanno positivamente vi saranno ragioni di ottimismo, anzitutto sul quadro libanese, il che ovviamente è indispensabile. Per quanto riguarda l'impegno politico dell'Italia - ed è la parte conclusiva del mio intervento noi ovviamente continuiamo l'azione a sostegno del dialogo. Abbiamo plaudito all'elezione di Sleiman ed abbiamo plaudito all'accordo di Doha, che era l'unica possibilità per far ripartire il Libano. Siamo all'inizio di una strada, non alla fine, ma è evidente che l'Italia è considerata in Libano con autorevolezza e prestigio: non abbiamo secondi fini; non abbiamo un passato se non di amicizia e di vicinanza e dobbiamo lavorare per contribuire alla stabilità di quel Paese. Ho rinnovato al presidente Sleiman il sostegno del Governo italiano al popolo e al Governo libanese e l'auspicio che il Governo si formi presto e che si possa dare respiro a quello che oggi è il nodo vero: stabilità e sicurezza da un lato, rilancio economico dall'altro. Ho anche colto l'occasione per confermare, come aveva fatto il ministro La Russa pochi giorni prima, il nostro sostegno alla missione UNIFIL 2. È una missione che, lo sapete già, riscuote apprezzamento unanime; ha garantito la realizzazione di una zona cuscinetto a Sud del fiume Litani. La risoluzione n. 1701

sempre secondo il mandato, spetta alle sole autorità libanesi il disarmo forzoso delle milizie sul terreno. È evidente che dobbiamo lavorare molto su questo aspetto:

Credo che una stabilizzazione definitiva - ad esempio, all'interno dell'auspicabile negoziato Israele-Libano, che dovrebbe portare a trasformare il cessate il fuoco in un cessate il fuoco definitivo - sarebbe un elemento fondamentale anche per contribuire alla sicurezza dello Stato di Israele. Si è molto parlato delle regole d'ingaggio: la lettura

per assicurare che quell'area di operazioni non sia utilizzata per attività ostili, non sia terreno di transito di gruppi armati o non sia usata per resistere alle missioni di UNIFIL. L'obiettivo su cui il ministro La Russa ha attirato recentemente l'attenzione è quello di applicare in modo efficace le regole che ci sono per la zona cuscinetto, il che vuol dire potenziare le attività congiunte con le forze armate libanesi, moltiplicare gli interventi di ispezione e controllo sul terreno. Vi posso dare alcune cifre: dopo la creazione di *check-points* congiunti tra forze libanesi e forze UNIFIL,

la nostra presenza a beneficio della popolazione libanese. In tutto questo, noi ci terremo strettamente in contatto con l'Europa,

la responsabilità che gli è stata assegnata con un'amplissima maggioranza sia riposta in un uomo che ha grandi capacità, almeno per quello che ho potuto valutare. Credo che sia anche importante che a questo evento abbia partecipato una foltissima delegazione della comunità internazionale; lei, signor Ministro, ha ricordato gli elementi di maggiore spicco, quelli che evidenziano le possibilità di relazioni future, ma io credo che sia stata importante proprio una partecipazione forte e corale. Tutti siamo soddisfatti degli accordi raggiunti, del fatto che si sia giunti all'elezione del Presidente, ma non sfugge a nessuno, e anche lei nella relazione lo ha sottolineato, che gli elementi di fragilità e di difficoltà sono ancora tutti presenti: lei ha citato la questione delle fattorie di Shebaa, ma c'è anche il problema dei militari israeliani ancora prigionieri, nonché le questioni che riguardano il processo Hariri, quindi il tribunale internazionale. Di fatto tutti gli elementi di tensione, compresi quelli che avevano portato alla crisi precedente (quindi il rapporto tra maggioranza ed opposizione e il potere di veto che adesso è stato concesso), rendono la situazione ancora terribilmente terribilmente fragile ed incerta. Si è aperta una finestra positiva in un momento in cui poteva precipitare la situazione; ovviamente ciò è motivo di soddisfazione per tutti.

Nel momento della campagna elettorale e della propaganda si può anche fare, ma penso che adesso sia il momento di passare a un dialogo più costruttivo.

per certi versi positiva, considerato il rafforzamento dell'autorità dello Stato sull'intero territorio, la riaffermazione precettiva di questo principio e l'impegno delle parti a non ricorrere all'uso della forza per finalità di carattere politico, nonché per la larga maggioranza che ha eletto il Presidente dello Stato. Per altri versi, però, è una fase ricca di aspetti problematici, come lei ricordava: tra questi, la questione della minoranza di blocco del futuro Governo di unità nazionale, con una sorta di sterilizzazione, quindi, anche del ruolo istituzionale di garanzia del Capo dello Stato, posto che i suoi tre Ministri i suoi tre Ministri avranno una funzione ridotta rispetto al passato (negli Esecutivi precedenti i tre Ministri avevano infatti una funzione per così dire di equilibrio, di garanzia, di moderazione e di mediazione tra la maggioranza e l'opposizione). Vi è poi il tema della legge elettorale

rende di fatto impossibile, sia all'ONU che all'UNIFIL, di prendere il controllo delle fattorie di Shebaa e degli altri territori occupati dagli israeliani.

riferimento che, di fatto, può essere vulnerato dal materiale possesso e dalla detenzione delle armi da parte di Hezbollah. Vi è poi un'altra questione, peraltro sollevata nella passata legislatura qui in Senato con un ordine del giorno - credo approvato il 27 marzo 2007 - con primo firmatario il collega Mantica,

Grazie all'applicazione integrale degli Accordi di Taif del 1989 e delle risoluzioni nn. 1559 e 1680, tendenti al totale disarmo dei gruppi che operano in Libano. È quindi necessario continuare su questa strada per porre fine alle interferenze siriane ed iraniane in quell'area e per garantire l'integrale ritiro di Israele da quei territori. territori. Signor Ministro, noi siamo qui a dirle che saremo vicini al Governo nell'azione che ha già intrapreso e che continuerà ad intraprendere, se proseguirà sulla strada che fino a qui ha tracciato; da parte nostra l'apprezzamento non è solo formale, quindi, ma è sostanziale di condivisione di un'azione. Le facciamo tanti auguri perché questa azione possa proseguire al meglio, nell'interesse anche del nostro Paese.

abbiamo ascoltato con molta attenzione le considerazioni e le valutazioni espresse questa mattina. La vicenda fu già all'attenzione del Senato all'indomani del conflitto dell'estate del 2006. Proprio in Senato si trovò una convergenza sulla partecipazione italiana a quello strumento, voluto dalle Nazioni Unite, che aveva dettato la fine delle ostilità. Nondimeno non mancarono in quella occasione tutta una serie di precisazioni e di distinguo. Ricordo, in particolare, le preoccupazioni - ahimè, molto fondate - espresse in quella occasione dal senatore presidente Marcello Pera. In questi due anni la situazione non è affatto migliorata. Quelle preoccupazioni del collega Pera, a proposito di un combinato disporsi di Hezbollah di città e di Hezbollah di campagna, anzi di montagna, tra il fiume Litani e i nostri soldati hanno costituito in qualche modo l'elemento di pressione che ha prodotto gli avvenimenti di cui questa mattina lei ha tracciato una nitida cronaca. Non Non c'è dubbio che è il momento nel quale bisogna avere anche una certa serenità nella garanzia di di neutralità, indipendenza e autonomia di quel martoriato Paese. Da questo punto di vista possiamo segnalare con soddisfazione l'iniziativa diplomatica degli ultimi giorni, che ha visto alcuni grandi Paesi europei finalmente a fianco e non a dispetto degli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America. Molti colleghi si sono già richiamati ad un più forte profilo europeo. Non saremo noi del Popolo della Libertà ad ostacolarlo. Però attenzione: non confondiamo, come avemmo la sensazione che molti facessero due anni fa, per politica europea la vecchia politica francese in Libano. Sono cose, vicende e tempi diversi. Per quanto riguarda la prospettiva di migliori rapporti, tramite la Turchia, tra la Siria ed Israele non abbiamo alcunché da eccepire: abbiamo soltanto da rimpiangere il velleitarismo con il quale certe volte la parte della Turchia, del facilitatore, l'hanno voluta fare alcuni esponenti del Governo precedente. Sotto questo profilo, onorevole Ministro, lei è già stato ministro degli affari esteri in un Governo Berlusconi e, mi pare quattro anni fa, ha avuto il merito di sollevare, proporre ed imporre ad un'Europa abbastanza recalcitrante l'inserimento di Hamas nella lista delle organizzazioni terroristiche. Non abbiamo quindi considerazione prudenziale in questo Parlamento, con ai banchi del Governo un Ministro come lei, per segnalare quanto poco giovino alla stabilità del Medio Oriente formazioni politiche

esattamente l'inverso di una norma della nostra Carta costituzionale. La definizione che viene usata di solito è Stati nello Stato, non già con riferimento al lessico della terza internazionale, dei partiti comunisti negli Stati di democrazia liberale, ma Stati, in questo caso la Siria e l'Iran, rispetto al martoriato Libano. Libano. Sappiamo anche che lei è un Ministro di fortissima sensibilità a quel capitolo di amicizia e simpatia con lo Stato di Israele che ha esaurito tutto il programma di politica estera del Presidente del Consiglio alle Camere. In nome di questi sentimenti sappiamo benissimo che quanti hanno plaudito alla grandezza d'animo dello scrittore israeliano Grossman, che è stato in Italia recentemente ed ha parlato senza odio di pace pur avendo perso un figlio in quella guerra di due anni fa, non dimenticano che il "fuoco nemico" che lo uccise era fuoco Hezbollah. Di qui tutta una serie di preoccupazioni implicite e sottese al suo intervento di questa mattina per il quale il Popolo della Libertà non può che formulare sentito apprezzamento.

numerosi incontri ai vari livelli che hanno contributo negli ultimi mesi all'uscita dalla crisi in Libano con il raggiungimento di un accordo globale caratterizzato dal prevalere di una rinnovata atmosfera di dialogo e di responsabilità del Paese non fanno altro che rinnovare l'attenzione sulla complessità e, talvolta, la precarietà degli equilibri interni ed esterni esistenti in quello scacchiere. L'annuncio di tale accordo il 21 maggio scorso, a margine di un vertice a Doha che, sotto la congiunta supervisione dell'emiro del Qatar, al-Thani, e del segretario generale della Lega araba, Amr Moussa, ha visto la partecipazione di numerosi Ministri degli esteri dei Paesi arabi, deve essere salutato come una tappa essenziale per la rimessa in funzione del sistema istituzionale. Esso ha dato un frutto immediato con la elezione, dopo circa sei mesi di voto istituzionale, del nuovo Presidente dello Stato libanese nella persona del generale Michel Sleiman in un ambito caratterizzato da ampio consenso e rinnovato spirito di ricerca di mediazione tra gli attori in gioco. Mi sembra in questo contesto - e lei lo ha citato - importante ricordare l'incontro informale sul Libano a Kuwait City il 20 aprile scorso che ha portato ad una dichiarazione degli "Amici del Libano". incontro che tanto informale non è stato visto che, come lei ha citato, erano presenti Ministri degli esteri ed inviati di Francia, Germania, Arabia Saudita, Egitto, Stati Uniti, Italia, Giordania, Kuwait, Qatar e Regno Unito con la supervisione del sempre presente e attento Amr Moussa, del Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e del Segretario generale delle Nazioni Unite. Dopo tre anni dal ritiro delle truppe siriane forse è il caso di auspicare che Siria e Libano possano normalizzare i loro rapporti nel mutuo rispetto delle sovranità territoriali e della indipendenza politica. Forse l'Italia può adoperarsi più concretamente affinché i due Paesi stabiliscano relazioni diplomatiche piene, delimitino la loro frontiera comune comune e rafforzino l'impegno a non consentire che il territorio dell'uno diventi terreno di azioni per destabilizzare l'altro. Signor Ministro, la partita che si gioca qui in Libano - è chiaro a tutti - non riguarda solamente il destino del Libano come Paese che uscì faticosamente da una disastrosa guerra civile ma la vicenda stessa dei Paesi dell'Asia centrale e del Mediterraneo, area a cui l'Italia annette in maniera spesso enunciativa noi diciamo sostantiva - prioritaria importanza per i suoi interessi politici, strategici, economici e culturali. È in questa fase raccomandabile massimo pragmatismo e massimo dispiegamento delle capacità proprie di promuovere un dialogo costruttivo, caratteristiche riconosciute all'Italia dalla comunità internazionale. Questo non solo verso la Siria, ma anche con l'Iran ed Israele proprio ora che si abbozzano timide prove di dialogo israelo-siriano e che in Iran sono in atto dinamiche che potrebbero portare il prossimo anno alla elezione come Presidente della Repubblica di un moderato (forse proprio l'attuale sindaco di Teheran). Colgo l'occasione per rammentare che l'Italia è sempre stata per l'Iran un interlocutore ricercato ed ascoltato ma essa, per motivi non sempre chiari, si è più volte sottratta a questo onore-onere. E' noto, ad esempio, come nella gravosa questione del conflitto congelato tra Armenia e Azerbaijan i due contendenti abbiano più volte ed in maniera neanche riservata dichiarato che l'Italia sarebbe un mediatore bene accettato da ambo le parti. A questo potenziale di mediazione il nostro Paese si è spesso sottratto, e non solo per i ben noti equilibri di politica internazionale. Lo spazio di azione per la comunità internazionale, per l'Unione europea e per l'Italia dipende anche molto dal coraggio e dall'autorevolezza del Governo che si instaurerà, che fermamente appoggeremo, insieme all'operato di tutte le altre forze istituzionali: la Presidenza che è stata appena ristabilita, il Parlamento, le Forze armate ed i Servizi di sicurezza. Così come abbiamo appoggiato tutti gli sforzi dell'attuale Governo, ora Governo di transizione, di Fouad Siniora. È di tutta evidenza però, signor Ministro, che solo l'autorevolezza e la compattezza istituzionale potrebbero permettere al nuovo Governo di dichiarare Hezbollah - il sedicente Partito di Dio - una forza illegale che si colloca al di fuori degli interessi di tutte le comunità del Libano e dei normali metodi che caratterizzano la dinamica di un Paese democratico. Senza questo passo coraggioso la comunità occidentale poco o nulla può fare per adoperarsi

Né sembra utile in questa fase interessarsi unilateralmente delle cosiddette regole di ingaggio, anche se la preoccupazione per l'integrità, la sicurezza e l'efficienza delle nostre truppe in Libano è sicuramente atto dovuto e lodevole. Ricordo che l'Italia è in Libano sotto l'egida e su mandato delle Nazioni Unite, insieme a forze di altri Paesi, un eventuale cambiamento delle regole operative che consentono di reagire alla minaccia - il cui grado negli ultimi mesi aveva raggiunto livelli sensibili di preoccupazione - può solo essere frutto di coordinamento e di concertazione con tutti gli altri partner. La scelta di nominare 16 Ministri espressi dalla maggioranza, 11 dalla minoranza e 3 dal Presidente è un buon viatico, ma la pietra angolare sarebbe quella di abbandonare, mano a mano, il rispetto della etnicità nella scelta ed assegnazione delle cariche, per optare verso elementi selezionati per la neutralità e le competenze specifiche. Sappiamo essere questo un passo difficile e comprendiamo che richiede la necessaria gradualità. Ma qui mi preme sottolineare, signor Ministro, un terzo aspetto operativo che riguarda il ruolo dell'Italia in Libano: si tratta della nostra missione più importante. Abbiamo la *leadership* della leva militare, ci troviamo nell'area del Mediterraneo, in un Paese dove sono presenti oltre 18 principali confessioni religiose e circa 26 diverse sfumature etniche; godiamo di un prestigio enorme e siamo sotto l'osservazione diretta di tutti gli interlocutori del bacino arabo e di quelli internazionali. Non possiamo, signor Ministro, commettere errori e non possiamo non giocare un ruolo di primo piano. o meglio di ripartenza, dopo l'insediamento del Presidente dello Stato libanese, è quello di riprendere lo spirito dei sette punti elencati già nel luglio 2006 dal primo ministro Siniora, che si basa sugli Accordi di che riconoscevano a mo' di compromesso la presenza e la funzione provvisoria di pacificazione delle truppe siriane in Libano, e sull'insieme delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (per la precisione le risoluzioni nn. 1559, 1680, 1701 e 1757), insieme alla sopra ricordata messa in opera delle iniziative della Lega araba. L'accordo, appena realizzato e sulla cui tenuta occorrerà vegliare attentamente, si ispira fortemente agli sforzi comuni di Italia, Francia e Spagna ed ai princìpi che già nel luglio 2007, in una riunione con i rappresentanti dei principali partiti libanesi, il suo collega francese aveva organizzato a Celle-Saint-Cloud. Il cammino e il ruolo che le Nazioni europee "mediterranee" da allora avevano avviato hanno certamente contribuito a portare sino al risultato di Doha. Anche una Nazione europea non mediterranea, ma straordinariamente attiva in quello scacchiere, la Germania, per bocca del suo Ministro degli esteri, ha assicurato un concreto supporto economico, logistico e politico al ristabilimento completo, e non ambiguo, dell'unità, della stabilità e della indipendenza del Libano. La valle della Bekaa dovrà tornare ad essere il polmone verde ed agricolo del Paese e non un corridoio, un varco per scorribande di agenti che esercitano una tutela extranazionale su un Paese la cui sovranità era fortemente ammalata. La crisi con Israele del 2006, lo ha ricordato lei, signor Ministro, è costata oltre 1.200 vite umane e danni stimati dal Governo libanese in oltre 3,5 miliardi di dollari; il successivo Summit G8 a San Pietroburgo e le due conferenze dei donatori nel dei donatori nel biennio 2006 e 2007, tenutesi a Stoccolma ed a Parigi, hanno permesso di reperire fondi per circa 8,8 miliardi di dollari da devolvere a sostegno della ripresa e della ricostruzione in Libano, a partire dalle donazioni di oltre 38 Stati. Concludo, signor Presidente, dicendo che questo è dunque un *turning point* della vita politica libanese ed un test essenziale per verificare se le forze all'interno del Paese e la comunità internazionale vicina al Libano siano in grado di scongiurare un peggioramento della situazione, che costituirebbe una deriva quasi certa verso uno stato di guerra civile, e di riavviare tutte le dinamiche politiche, istituzionali, economiche, sociali e culturali che l'Italia sostiene con piena forza sia come agente di politica internazionale presente in modo diretto ed indiretto sul teatro libanese, che come soggetto tutelante i propri interessi ed il proprio prestigio nell'area centro-asiatica e del bacino mediterraneo. Facciamo dunque gli auguri per questa grande missione che abbiamo davanti, ma come diceva la collega del Partito Democratico che mi ha preceduto, dobbiamo farlo tutti insieme con senso di responsabilità per il nostro Paese e per l'immagine che daremo

la sicurezza dei nostri soldati. Voi avete in mano le leve, gli strumenti, le regole di ingaggio, che sappiamo non essere materia da disciplinare in Aula in modo legislativo, ma è anche vero che possiamo rivolgere al Governo un invito senso. Se a livello UNIFIL esistono regole comuni, dobbiamo sapere anche che in Afghanistan non abbiamo le stesse regole

Ministro, abbiamo appreso da quotidiani israeliani, come "Haaretz", che non gradiscono molto la nostra presenza un tantino

una presenza che oggi può apparire quasi paradossale. Accade questo,

i sobborghi sciiti di Beirut ovest, ha fatto incursioni in sedi televisive appartenenti a partiti contrapposti; il figlio di Hariri ha fatto chiudere addirittura un giornale

Fonti ONU ci dicono viceversa che sulla cortina tra il fiume Litani e il confine israeliano la situazione è del tutto pacifica. Noi e i Caschi blu stiamo presidiando la zona,

Possiamo far finta di nulla, ma ormai anche i rotocalchi ci danno le notizie di cosa avviene: dalla Siria passa di tutto; arrivano sul confine israeliano armi di produzione russa, dall'Iran arrivano altri aiuti. Ministro, noi dovremmo dire una cosa: probabilmente in questo frangente è molto più importante un'azione diplomatica che rafforzare rafforzare o decuplicare un contingente che si troverebbe sempre in condizioni di difficoltà, soprattutto in un contesto estremamente difficile e del tutto avverso.

e noi pensiamo che forse abbia svolto più lavoro all'estero che non nel suo ufficio che probabilmente non sarà nemmeno ultimato e non avrà potuto ancora vedere funzionante. come Gruppo della Lega Nord, caro Ministro, la prima nostra esigenza: abbiamo a cuore che il Mediterraneo sia il più pacifico possibile. È un po' la nostra trincea; se non vi fosse stata quell'area, probabilmente avremmo spostato verso di noi tante più tensioni e conflitti, però, in questo momento noi le raccomandiamo la massima sicurezza per i nostri militari

si racconta quel che succede quasi fossimo fatti dalle cose, senza mai analizzare come si arriva a costruire quelle cose. Ci ha descritto quello che è successo e ci ha ricordato che sono state ammazzate 72 persone soltanto nel mese di maggio e almeno una mezza dozzina di parlamentari della maggioranza, che ci sono quasi mille feriti soltanto negli ultimi mesi, ma non ci sono stati dati un giudizio o un'analisi politica da parte sua e da parte del Governo Berlusconi sul modo in cui si è arrivati a dare alla Lega araba (la lega di Stati non democratici) il potere di giungere a un compromesso. Dico questo perché - é stato ricordato poco fa la parte conclusiva dell'intervento del presidente Berlusconi alla Camera, quando ha chiesto la fiducia, si è incentrata tutta sulla necessità di garantire la sicurezza a Israele. Una delle prime dichiarazioni che il presidente Sleiman ha fatto é stata quella

La prospettiva per cui 11 Ministri su 30 saranno del blocco che fa riferimento ad Hezbollah - che sicuramente è un partito politico, ma che ha anche delle fazioni militari armate che sono state la causa della guerra del 2006 non credo vada necessariamente nella direzione auspicata dal presidente Berlusconi di difesa dello Stato d'Israele. Ancora più preoccupante in quel che lei ci ha detto oggi è che due sono, secondo lei, gli elementi che trova ulteriormente positivi rispetto agli Accordi di Doha: la stabilità da una parte e la sovranità dall'altra. Ecco, non credo che nel 2008 la sovranità assoluta di uno Stato Nazione possa, in qualche modo, concorrere non soltanto a trovare la pace - che non è mai apparsa nel suo discorso -, ma neanche la stabilità. Quindi, c'è bisogno di recuperare un'iniziativa politica ben precisa e non soltanto diplomatica e militare, per quanto anche queste siano assolutamente necessarie. Il gruppo degli «Amici del Libano» deve essere composto dagli Stati membri dell'Unione Europea per ampliare

Due sono i punti fondamentali, a mio parere estremamente positivi, fermo restando che concordo con i pro e i contro da lei elencati. Il primo punto è che Hezbollah ha accettato questo discorso. Chiunque abbia una minima conoscenza dell'ambiente libanese sa che Hezbollah condizionava sempre in maniera estremamente negativa le parole di Siniora, di Hariri e di

sia già in trattativa con Israele, come da lei affermato con una certa serietà, a mio parere è molto importante e di grande rilievo per la stabilità. Se ho

vorrei aggiungere che, come precedentemente comunicato ai Gruppi per le vie brevi, all'inizio della seduta pomeridiana di oggi ricorderemo il cinquantesimo anniversario di attività parlamentare del senatore Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica.